nei confronti di Carlo Maria Maggi e di Maurizio Tramonte, riconoscendoli colpevoli della efferata strage consumata in piazza della Loggia, nella mia città, il 28 maggio 1974, quarantatre anni fa. Prendo la parola con una qualche emozione perché penso che, finalmente, gli amici e i compagni che sono morti vittime della strage di piazza della Loggia possono riposare in pace. Parlo di amici e compagni perché intrattenevo una frequentazione diretta e personale con molti di loro. Amici e compagni, perché non uso, come fanno altri, la parola compagno come una clava contundente, credo che dica di una storia e di una biografia. Per me anche questa sentenza costituisce una sorta di liberazione. Da sindaco della città ho vissuto tutto il travaglio di una dolorosissima assenza di verità e sento anzitutto di portare la mia solidarietà al nostro collega, parlamentare in carica, onorevole Alfredo Bazoli, la cui madre è caduta in piazza della Loggia. Quali considerazioni si possono trarre da questa vicenda? Sono passati e soltanto dopo una storia fatta di reticenze, omissioni, depistaggi e menzogne, finalmente assistiamo a un'effettiva sovrapposizione fra la verità storica, che era ormai acquisita, e quella giudiziaria. acquisita, e quella giudiziaria. Nel 1994 ho invitato uno dei buoni maestri del pensiero politico italiano, Norberto Bobbio, a sviluppare una riflessione sul tema della memoria. Ebbene, in quella straordinaria occasione il filosofo teorizzò un rapporto strettissimo tra la verità e la giustizia: finalmente abbiamo giustizia perché abbiamo verità e abbiamo verità perché abbiamo giustizia. Questa verità dice di un intreccio perverso e di una cospirazione promossa da soggetti e movimenti che fanno riferimento al radicalismo della destra estrema e anticostituzionale e a settori e apparati dello Stato assolutamente infedeli alla Costituzione. Ma questa storia documenta e testimonia anche di un impegno assunto da uomini delle istituzioni, magistrati, esponenti politici,

perché lì vi è stato un elemento straordinario di tenacia civile da parte delle forze democratiche e dei familiari delle vittime, delle vittime, che hanno saputo andare contro tutto quello che poteva apparire il mondo e, soprattutto, lo Stato italiano nei suoi corpi più delicati

alla sentenza e alla condanna, certo di due soli colpevoli in vita.

con organizzazioni eversive volte a colpire le istituzioni e le associazioni della democrazia, i partiti di sinistra, il movimento sindacale. No.

non si è saputo prendere alcun provvedimento cautelare. Parlo persino di quelli più banali, come il divieto di espatrio e,il ritiro del passaporto; tant'è che poche ore fa uno dei due condannati all'ergastolo, Maurizio Tramonte, è stato arrestato in Portogallo presso la località di Fatima. Questo ci squaderna una responsabilità che non voglio pensare come in quegli anni, con la doppiezza e la servitù degli apparati dello Stato a organizzazioni illegali, clandestine e, eversive; ma di certo ci dice che dobbiamo fare quello che non è stato fatto e che c'è tutto da fare. La catena va interrotta, quella che, poche ore dopo la strage, diede l'ordine al comando dei Vigili del fuoco di pulire la piazza con le pompe idrauliche, per non avere più la possibilità di indizi di qualsiasi tipo, prima ancora che intervenisse la magistratura. Ecco, credo che, davvero, se vogliamo onorare le vittime e i familiari di tutte le tante, troppe vittime delle terribili stragi che hanno costellato quegli anni,

violento nei confronti di qualsiasi consesso sociale e associazione che può promuovere attività e manifestazioni, che non possa accadere mai più che i maggiori vertici del nostro Stato siano non solo collusi, ma facciano parte direttamente e, scientemente,

Sì, perché Maurizio Tramonte era un informatore a libro paga dei nostri Servizi. Ecco, credo che dobbiamo dire «mai più!» in maniera non retorica, con l'impegno di oggi e per il futuro.

dare notizia e commentare la sentenza della Corte di cassazione che ieri ha confermato la pena dell'ergastolo per due dei responsabili della strage di piazza della Loggia a Brescia, confermando così le condanne emesse nel secondo processo d'appello del 22 luglio 2015 nei confronti di Carlo Maria Maggi, ai tempi capo di Ordine Nuovo nel Veneto, e di Maurizio Tramonte, iscritto nel 1973 a libro paga dei Servizi segreti dello Stato. Due ergastoli, con uno dei condannati già in fuga ieri, ma per fortuna assicurato dalle Forze dell'ordine alla giustizia e al carcere. carcere. Vorrei ricordare quanto accaduto quella lontana, lontanissima mattina del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia a Brescia: erano tantissimi i cittadini riuniti per una manifestazione antifascista, una manifestazione pacifica indetta dai sindacati e dal Comitato antifascista per protestare contro la violenza neofascista che in quei giorni e in quei mesi stava interessando il Paese. Una bomba nascosta in un cestino, fatta esplodere mentre era in corso la manifestazione, provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre In quella stessa piazza, occorre ricordarlo, il 25 aprile 1969 era stata fatta saltare la lapide dedicata ai partigiani che avevano sacrificato la loro vita nella lotta contro il nazifascismo e per la liberazione del nostro Paese. In quello stesso 25 aprile, dedicato a celebrare la resistenza e la liberazione dell'Italia, sempre a Brescia venne devastata la sede dell'Associazione nazionale partigiani. In quel 1969 vi furono in Italia ben centoquarantacinque attentati dinamitardi, in gran parte di matrice neofascista. Fu un anno tragico, che culminò il 12 dicembre 1969 con la strage di piazza Fontana a Milano, che causò la morte di sedici persone e il ferimento di altre ottantaquattro. Iniziava così un periodo cupo per la nostra Repubblica. Più di un decennio di violenza e di terrore: da piazza Fontana alla strage di Peteano del 31 maggio 1972, poi la strage del treno Italicus il 4 agosto 1974, con dodici morti fino alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 con ottantacinque morti e duecento feriti. Una lunga scia di sangue e di terrore, con centinaia di morti e feriti, per la quale, fino a ieri, non c'erano colpevoli, tante, troppe, stragi impunite. Ora, la sentenza ci consegna finalmente una verità giudiziaria ufficiale e definitiva e con essa la conferma di una verità oramai conclamata sul piano storico. La strage e il suo movente si iscrivono a pieno titolo all'interno di un disegno eversivo più grande, quello della strategia della tensione, che ha condizionato per oltre un decennio la vita della nostra Repubblica e con essa la nostra vita. Una sentenza straordinariamente importante, quindi, perché si tratta del primo attentato ad essere qualificato giuridicamente come strage politica e il peculiare contesto in cui venne realizzato non lasca adito a dubbi sulla connotazione e matrice, come è scritto nella sentenza della corte d'appello ora confermata in Cassazione. La sentenza chiarisce, quindi, in modo irrevocabile che l'attentato di piazza della Loggia è maturato nello stesso ambiente delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe tra il 1969 e il 1980. L'individuazione dei due responsabili rappresenta emblematicamente il grave e tragico connubio fra la destra eversiva e pezzi deviati di apparati dello Stato. D'altra parte, dopo cinque istruttorie e 13 dibattimenti, dopo proscioglimenti e assoluzioni, proprio il lungo processo, porta una traccia, cosi è scritto nella sentenza, dell'«opera sotterranea portata avanti con pervicacia da un coacervo di forze individuabili in una parte degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, dai servizi americani alla P2, che hanno prima incoraggiato e supportato lo sviluppo di progetti eversivi della destra estrema e poi hanno sviato l'intervento della magistratura rendendo di fatto impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità». In una riflessione su quegli anni, Aldo Moro affidò al suo Memoriale queste parole: la cosiddetta strategia della tensione ebbe la finalità, anche se fortunatamente non conseguì il suo obiettivo, di rimettere l'Italia nei binari della "normalità " dopo le vicende del '68 e dell'autunno caldo. «È doveroso alla fine rivelare che quello della strategia della tensione» così continua Aldo Moro nel memoriale «fu un periodo di autentica e alta pericolosità, con il rischio di una deviazione costituzionale che la vigilanza delle masse popolari non permise». Si trattò, come sappiamo, di spinte eversive accomunate dall'obiettivo di ostacolare l'avanzata di forze innovative, sia in ambito politico che in ambito sociale.

Una lunga scia di terrore e di sangue, una storia che occorre insegnare ai giovani; la maggior parte di loro non conosce infatti le vicende tragiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese negli anni Settanta, con lo stragismo di matrice fascista.

che vengono condannati due responsabili di una strage politica. Insieme alla soddisfazione per questa sentenza, certamente, rimane l'amarezza e un grande rammarico per un verdetto che arriva dopo quarantatre anni, molto tardi, troppo tardi per dare la giusta punizione agli altri responsabili di quella strage, perché oramai non ci sono più. Infine, vorrei esprimere un sentimento di vicinanza e un ringraziamento a quanti, magistrati, investigatori, istituzioni e cittadini, hanno consentito di arrivare a questa sentenza. In particolare, vorrei esprimere, a nome del Gruppo del Partito Democratico, un sentito ringraziamento all'Associazione dei familiari delle vittime, che non si è mai arresa e che instancabilmente, in questi lunghi decenni, ha chiesto verità e giustizia. Verità e giustizia che finalmente ora abbiamo, almeno per la strage di piazza della Loggia, e che erano dovuti innanzitutto alle vittime innocenti, ai loro familiari, alla città di Brescia e, con essa, a tutto il nostro Paese.

al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate",

Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione pregiudiziale QP1 e la questione sospensiva QS1.

Vi chiedo un attimo di attenzione, perché è una questione che viene da noi sollevata, nonostante non abbiamo presentato emendamenti in Commissione, né abbiamo fatto ostruzionismo

che pone in discussione la serietà del nostro Parlamento nell'affrontare i problemi di mafia. Nella seduta del 13 giugno ultimo scorso, a seguito di un dibattito riguardante la mancata espressione da parte della 5ª Commissione del parere sul provvedimento in titolo, nel quale sono intervenuti il Presidente, il rappresentante del Governo e alcuni senatori esponenti dei vari Gruppi, la medesima Commissione, su proposta del correlatore, ha deliberato a maggioranza di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta successiva. Nella medesima seduta, come già avvenuto in una precedente convocazione del 1° giugno, il Presidente della Commissione ha ribadito: «La Commissione ha la possibilità di conferire il mandato ai relatori, relatori, pure in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1° giugno 2017 la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno, sul presupposto che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5a Commissione, occorre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il parere predetto non dovesse arrivare entro oggi». A tale riguardo ha sottoposto la questione alla valutazione dei membri della Commissione. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Migliore, ha dichiarato che il vice ministro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio sulla necessità di definire soltanto alcuni aspetti tecnici, evidenziando che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe fatto pervenire, nel corso della stessa giornata, una nuova relazione, favorevole, sulla relazione tecnica presentata dal Ministero della giustizia, per consentire alla Commissione bilancio di esaminare ed infine approvare il parere. Su tale aspetto sono stati sollevati, da più parti, dubbi di carattere procedurale e sostanziale, ravvisandosi la necessità di condizionare il conferimento del mandato ai relatori alla previa acquisizione del parere della Commissione bilancio, ciò al fine di evitare che il testo potesse presentare significativi elementi di criticità rispetto al vincolo di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. A tal fine occorre richiamare, altresì, l'attenzione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di lunedì 12 giugno, di due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura finanziaria, i quali poi, in serata, sono stati ritirati dai relatori medesimi. Nella seduta del 14 giugno, il Presidente ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione, rilevando l'opportunità di apportare modifiche al testo approvato dalla Commissione, per recepire le condizioni imposte dalla Commissione bilancio, mediate presentazione da parte dei relatori di proposte di coordinamento

con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le citate modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale; come abbiamo osservato in Commissione, le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio non avrebbero potuto essere recepite mediante proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin a quel momento dalla Commissione giustizia; che regolano il procedimento legislativo, i relatori, per recepire le predette condizioni, avrebbero dovuto presentare ulteriori emendamenti rispetto ai quali di conseguenza avrebbe dovuto essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti; giova, inoltre, rilevare che, trattandosi di un provvedimento complesso e caratterizzato da un lungo *iter*, sarebbe stato preferibile *iter*, sarebbe stato preferibile allora votare il conferimento del mandato ai relatori senza recepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bilancio, rinviando al momento della discussione in Assemblea il recepimento delle stesse; per i motivi suesposti, tale *modus procedendi* reca una palese violazione dei principi basilari del procedimento legislativo, che espone il nuovo testo del codice antimafia al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale,

come, trattandosi di mafia, non vorrei consegnare agli avvocati dei processi di mafia un argomento per il blocco delle norme che andiamo ad approvare; non vorrei consegnare agli avvocati dei processi di mafia la possibilità di eccepire costituzionalmente, se fossi ancora magistrato, accoglierei le eccezioni di costituzionalità, tenuto conto delle decisioni già pervenute in altri procedimenti della Corte costituzionale. Per le stesse ragioni, appare arduo inquadrare le modifiche votate nella seduta del 14 giugno in un'opera di coordinamento, ravvisandosi in alcune di esse profili sostanziali, come la proposta di coordinamento 25.Coord.100, concernente la copertura delle spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Con riferimento alla proposta di coordinamento 25.Coord.200, richiamo l'attenzione sulle disposizioni in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 113-*bis,* introdotto dall'articolo 27 del disegno di legge, che dovrebbe essere attribuito all'Agenzia sulla base del principio della mobilità, previsione questa che esula dal principio di efficienza dell'Agenzia nella quale dovrebbe essere incardinato solo personale altamente qualificato. Giova rilevare ancora che la proposta di coordinamento 29.Coord.100 non ha i requisiti di un mero coordinamento di forma, ma di vera e propria modifica sostanziale, che si evince dall'alinea che indica un intervento sostitutivo dell'articolo 29 (ora articolo 32), recante la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Signor Presidente, nella questione pregiudiziale sospensiva viene anche accennato al problema della non facile soluzione della doppia competenza tra procuratore distrettuale e procuratore circondariale. Mi auguro - e qui richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e dell' intera Assemblea - che si voglia fare una riflessione seria su quello che ho appena detto, perché anziché

l'altra invece è più tecnica e attiene alla pregiudiziale di incostituzionalità. non tutti i provvedimenti, ancorché costituzionali, meritano il nostro apprezzamento.

quindi, conseguentemente, ci sarà un voto in linea con questa considerazione. Il tema della pregiudiziale, però, è un tema squisitamente tecnico. Si solleva Si solleva un dubbio di costituzionalità per una violazione dell'articolo 77 della Costituzione ovvero del regolare *iter* legislativo del provvedimento che stiamo esaminando. Il senatore Caliendo è un raffinato giurista e non sono certo io a potermi assumere l'autorità di dargli suggerimenti o indicazioni,

la sentenza n. 9 del 1959 e l'altra, molto più recente, n. 262 del 1998. In buona sostanza, che cosa ha detto la Corte in entrambe

un difetto nel procedimento e nell'*iter* legislativo che porta all'approvazione di una legge, non attiene alla competenza della Corte Corte costituzionale l'eventuale rilievo di incostituzionalità, in quanto alle Camere e al Parlamento è devoluto ogni giudizio e ogni rimedio avverso eventuali errori di procedimento. Il senatore Caliendo dice sono state presentate due proposte di coordinamento, che possono ben dirsi anche emendamenti, da parte dei relatori, per le quali andava dato un termine in Commissione per eventuali subemendamenti. La vicenda, tale e quale, è stata

la Corte costituzionale ebbe a ribadire il principio che già aveva espresso nel 1959, secondo il quale, seppure vi è una violazione nell'*iter* legislativo, nel percorso del procedimento del Parlamento, questa irregolarità essere risolta dalla Corte costituzionale. Detto ciò, è chiaro che la questione di incostituzionalità non c'è e non vi può essere, e non possiamo ancora disturbare la

Ciò premesso, rimane la questione di opportunità di rimandare in Commissione il provvedimento. Sul punto che cosa posso dire? Per quanto mi riguarda, il provvedimento è talmente sbagliato in tutto che, secondo me, anche tornando in Commissione non ci possono essere rimedi che possano rendere questo un prodotto un prodotto accettabile da parte nostra, degli italiani e dei giuristi. Basti semplicemente considerare che le misure di prevenzione vengono estese anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Faccio un esempio banale: per un peculato d'uso, cioè per aver utilizzato la macchina impropriamente da parte di un amministratore, ci può essere l'applicazione delle misure di prevenzione, cioè si deve ritirare la sera entro una certa ora si possono confiscare i suoi beni. Signori, questo è un prodotto che offende tutti gli operatori del diritto. Io mi rifiuto di pensare che ci possa essere un magistrato che dovrà applicare una misura di tal genere, perché obbligato dalla legge

difficoltà a fare provvedimenti che vanno in questa direzione e che - ahimè - saranno costretti a fare, perché c'è una norma che glielo impone. Io questa norma

alla questione di incostituzionalità, quello è altro tema, squisitamente tecnico. Ho detto e ripeto che non sempre tutto ciò che è costituzionale è bene ed è buono. Questo è costituzionale, ma non è buono.

fatta dal senatore Caliendo, delle questioni sospensiva e pregiudiziale, egli ha citato a memoria ben due sentenze della Corte costituzionale; e di questo non posso che compiacermi. Purtroppo dimentica la terza, terza, quella che ha sancito l'incostituzionalità della cosiddetta legge Giovanardi, proprio perché era stato violato il procedimento legislativo con riferimento all'omogeneità della materia su un decreto-legge. Detto questo, che mi consente solo per l'ennesima volta di congratularmi con il senatore Falanga, vengo al merito della questione, cioè all'ordine dei lavori, signor Presidente.

serie e tecnicamente non di facile lettura. il codice antimafia, il quale, al di là della pregressa attività, io sono particolarmente legato, perché ebbi l'onore di firmarlo da Ministro della giustizia. L'interesse che il senatore Caliendo, io e il Gruppo di Forza Italia abbiamo è quello di andare avanti con un provvedimento che non sia in alcun modo aggredibile in sede giudiziaria, evidentemente con riferimento alla Corte cioè stabilire, non con l'emozione e la velocità di una pratica burocratica, se effettivamente vi è stata o non vi è stata una violazione del procedimento legislativo. So bene che vi sono cinque precedenti che consentirebbero questo coordinamento formale, ma dico anche che, a fronte delle osservazioni e delle condizioni che normalmente vengono poste dalla Commissione bilancio, probabilmente cinque precedenti sono pochi per individuare una prassi. Quindi, signor Presidente, io credo che vi sia la necessità di un momento di riflessione, cioè sostanzialmente di andare al voto su tale questione consentendo a tutti quanti noi di studiarne, per chi lo vorrà fare, il merito, per poi poterci determinare nel modo migliore possibile. Non sarebbe una perdita di tempo, signor Presidente, perché, ove mai noi dovessimo sbagliare su questo, anzi su un articolo, il 32, e su un altro segmento, che riguardano in maniera specifica l'Agenzia per i beni confiscati. Uno strumento, cioè, che si sta cercando di potenziare proprio per rendere più effettivo ed efficace il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. quindi, di una ragione di tipo ostruzionistico, ma di una ragione di prudenza, tutta rapportata all'importanza del provvedimento Io non credo, signor Presidente, che che votare questa questione sospensiva oggi o votarla alla ripresa dei lavori martedì sia un forte cedimento da parte della maggioranza o sia una vittoria dell'opposizione. Credo che sia semplicemente la strada del buonsenso. Potrei dire, facendo forse l'esempio più eclatante, che si stabilisce una disciplina *ad hoc* per il tribunale di Trapani e per il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, evidentemente immaginando che siano le sedi

facendo riferimento a Castelvetrano, fa riferimento al tribunale di Marsala e non al tribunale di Trapani. Ma non lo voglio dire, signor Presidente, perché non mi interessa: mi interessa semplicemente che l'Assemblea dia un voto consapevole sul problema sollevato e lo dia con grande serietà e con grande serenità

di volersi determinare per un piccolo intervallo, così da consentire che il voto abbia luogo martedì alla ripresa dei lavori, un voto che ciascun darà come meglio riterrà, ma che sia un voto in cui ciascuno di noi abbia avuto la possibilità di conoscere e conseguentemente di assumere le proprie responsabilità in maniera consapevole

dei Regolamenti parlamentari sfuggono ad ogni controllo di costituzionalità. Per dirla usando un linguaggio di diritto costituzionale, non si tratta di norme interposte. Sul punto è quindi inutile intervenire ulteriormente, se non per sottolineare che non si capisce quale sia il ruolo dell'articolo 77 della Costituzione, secondo il quale il Governo non può emanare atti dotati di valore di legge se non in virtù di una delega

Vengo alla questione sospensiva e alle tante questioni che vi ruotano attorno. In questo caso sostanzialmente ci si lamenta del fatto che le condizioni imposte dalla 5a Commissione, ai ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione, siano state recepite ai sensi dell'articolo 103 del nostro Regolamento, quindi con emendamenti singolarmente votati dalla Commissione giustizia e che, al contrario, non si sia conferito, assegnato, un termine per subemendare le condizioni imposte dalla 5a Commissione.

sostanzialmente parificabili ad emendamenti e come tali subemendabili. Si affermerebbe cioè un principio, il quale ovviamente non può essere affermato per la evidente ragione che non si tratta di emendamenti, ma di condizioni, le quali oltre tutto devono essere recepite in funzione di un percorso di costituzionalità Il paradosso consiste proprio nella circostanza di aver sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento al recepimento di condizioni che, al contrario, rendono costituzionalmente conforme quel processo di attività legislativa. Non è infatti un caso - e cito il linguaggio della prassi parlamentare, che significa fonte del diritto parlamentare che gli emendamenti o proposte di coordinamento (perché in questo caso la differenza è soltanto nominalistica) che recepiscono le condizioni imposte dalla 5a Commissione vengano definite emendamenti necessari nell'attribuito di necessari c'è la circostanza che non si tratta di veri e propri emendamenti, cioè di interventi di modificazione del testo, ma di recepimenti volti all'adeguamento del testo a principi costituzionali di bilancio. È opportuno chiarire che non si è trattato di emendamenti dei relatori nel senso generalista del termine, ma per l'appunto di emendamenti votati singolarmente dalla Commissione giustizia. Passerò adesso alla norma regolamentare di riferimento, rispetto alla quale si è manifestata la volontà dei componenti della Commissione giustizia. Il *vulnus* che si sarebbe verificato nel caso in cui la Commissione non fosse stata chiamata a manifestare la sua volontà rispetto a questi strumenti che recepiscono le condizioni della 5a Commissione, al contrario si è manifestata attraverso l'esercizio del diritto di voto espresso con riferimento ai singoli emendamenti che sul punto sono stati presentati. Mi permetto di sottolineare, sia pur superfluamente (io mi rivolgo al Presidente, ma contestualmente a tutta l'Assemblea) che l'articolo 103 sotto la vigenza del quale questi emendamenti di recepimento sono stati votati, consente modificazioni sostanziali del testo, dal momento che in quella disposizione compare il riferimento alla necessità di correggere norme rivelatesi incompatibili o inconciliabili con gli scopi assegnati alla legge. Di talché si ha l'evidente manifestazione della portata sostanziale, non formale, delle modificazioni introducibili attraverso il sistema preveduto dall'articolo 103 del nostro Regolamento, che implica non il coordinamento formale, che i relatori compiono in virtù del mandato loro conferito a conclusione del processo legislativo che si svolge in Commissione. Quelle sono proposte di coordinamento formali. Questa è un'altra cosa. L'articolo 103 prevede delle proposte di coordinamento sostanziali perché, per l'appunto, nel rispetto del dato letterale dell'articolo 103, sono funzionali a rendere compatibile e conciliabile il testo legislativo con lo scopo attribuito alla legge. Quindi, è chiaro che, se si deve rendere compatibile ogni disposizione con le finalità assegnate alla legge, si ha un mandato davvero amplissimo alla modificazione sostanziale del testo. Ripeto, però, che questa modificazione sostanziale del testo qui non si è verificata perché la Commissione si è limitata, votando singolarmente gli emendamenti, a recepire quelle condizioni che rendono costituzionalmente conforme il testo. Signor Presidente, io mi sono permesso di fare riferimento alla prassi come fonte del diritto parlamentare. Ne ha parlato il presidente Palma e io sono costretto a farlo in maniera del tutto sintetica, perché noi annoveriamo un precedente della Commissione giustizia del 2015, che decide nel senso nel quale la Commissione ha ritenuto di decidere. Vi è poi un altro precedente del 2005, sempre della 2a Commissione, che, recependo le indicazioni della Commissione bilancio, procede ai sensi dell'articolo 103; un precedente del 2005 della 1a Commissione, un precedente del 2005 della 13a Commissione (gli atti, ovviamente, sono disponibili) e un precedente del 2004 della 7a Commissione.

in materia di disposizioni concernenti i collaboratori di giustizia. Seguendo la procedura di cui all'articolo 103, con approvazione, mediante votazione, dei singoli emendamenti, si è deciso nella correlativa seduta di introdurre una disposizione che estendeva le disposizioni, fino a quel momento dettate solo per i collaboratori di giustizia, anche ai testimoni di giustizia. Con un coordinamento, quindi, votato ai sensi dell'articolo 103, si è duplicata la portata della disposizione legislativa perché la si è estesa dai collaboratori anche ai testimoni di giustizia. Contestualmente, si è introdotta anche una ulteriore disposizione che rendeva applicabili quelle disposizioni non soltanto a coloro i quali fossero divenuti collaboratori di giustizia dopo l'entrata in vigore della legge, ma anche a coloro i quali lo fossero da prima. Nel contesto delle indicazioni che io ho il dovere di dare all'intera Assemblea ve ne è anche un'altra, che ricalca temi noti del diritto parlamentare sul versante della prassi. della eventuale approvazione delle condizioni poste dalla 5a Commissione, che all'epoca non erano neanche intervenute (parlo della data del 23 maggio), risulta dal Resoconto della seduta della Commissione giustizia del 23 maggio. Quindi, i signori senatori sono stati informati della indicazione che il Presidente si era permesso di fare, secondo la quale, allorquando fossero giunte le condizioni frapposte dalla Commissione bilancio, queste sarebbero state votate con le modalità dell'articolo 103 del Regolamento. In quel contesto nessuno ha sollevato alcuna obiezione. Cito la prassi parlamentare del *nemine contradicente* per segnalare la circostanza per cui, in quel contesto, nessuno dei presenti ha obiettato legittimando il ricorso a una procedura che era stata anticipata di tre settimane rispetto al momento in cui poi il problema si è posto. Infatti,

la rilevanza di un vizio procedurale è data dalla misura del pregiudizio che la violazione ha determinato. Non vi è ovviamente alcuna violazione al riguardo... Oltre alla violazione mancante di ogni principio, concorre una prassi parlamentare assolutamente...

Sulla questione procedurale sono intervenuti il senatore Falanga (su tutte e due le questioni) e, poi, il presidente della Commissione giustizia, senatore D'Ascola. Poi il senatore Sposetti evidentemente non è riuscito a seguire bene queste cose.

se il tema è far iniziare la discussione generale nella seduta di martedì pomeriggio, noi non abbiamo problemi.

la Presidenza osserva preliminarmente che la proposta di coordinamento costituisce un istituto che il Regolamento prevede per finalità di coerenza logico-formale del testo e per ovviare a eventuali errori materiali. Tuttavia, le proposte di coordinamento approvate in Commissione, pur essendo volte ad adeguare il testo alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, recano modifiche di carattere sostanziale che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti. Ciò premesso, però, va osservato come in Commissione le modalità di votazione delle proposte di coordinamento e degli emendamenti risultino del tutto identiche, non sussistendo la possibilità, prevista invece per l'esame in Assemblea, di richiedere per i soli emendamenti modalità aggravate di scrutinio. Ferma, quindi, la necessità di confermare la linearità procedurale fissata nel Regolamento per i lavori delle Commissioni, si può comunque rilevare che la possibilità di ricorrere a proposte di coordinamento era stata preannunciata dal Presidente della Commissione giustizia nella seduta del 23 maggio scorso, come ci ha appena ricordato, a seguito del protrarsi della mancata espressione del parere della 5a Commissione ben oltre i termini regolamentari previsti. In tale occasione, peraltro, come è stato ancora una volta ribadito, non si sono registrate obiezioni rispetto alla soluzione procedurale proposta. Sebbene la Presidenza intenda ribadire il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita, senza dubbio il procedimento in sede referente si configura come più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea. In punto di fatto, la presentazione di una serie di proposte di coordinamento di carattere estremamente puntuale, riferite ciascuna a singoli articoli o porzioni di testo, ha consentito un esame sufficientemente analitico in conformità ai principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni sanciti dall'articolo 102, comma 4, del Regolamento. Anche il rilievo, in ordine alla lamentata compressione della facoltà di presentare subemendamenti determinata dalla scelta di ricorrere allo strumento della proposta di coordinamento non sembra, tuttavia, tuttavia, implicare conseguenze di rilievo sotto il profilo del rispetto dei diritti garantiti a ciascun parlamentare. La formulazione letterale dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, consente infatti a ciascun senatore la presentazione di proposte di coordinamento alternative. La possibilità di intervenire nuovamente sul testo della Commissione attraverso la presentazione di ulteriori proposte di modifica resta in ogni caso pienamente garantita dal successivo esame in Assemblea, come dimostrano gli emendamenti già presentati dai senatori Caliendo e Palma, volti a ripristinare in diversi passaggi il testo originario approvato dalla Camera dei deputati. Alla luce di tali considerazioni, in forza dei principi di conservazione degli atti e di economia procedurale, fermo restando che quanto accaduto non può comunque costituire precedente, la Presidenza ritiene di poter proseguire l'esame del provvedimento. Questo è quanto ha deciso la

A me dispiace, senatore Sposetti, ma - devo dire la verità - non costringo nessuno ad ascoltarmi.

In un passaggio del suo discorso, lei dice che sarebbe stato preferibile fare degli emendamenti, ma sostanzialmente, essendo state votate le singole proposte di coordinamento, alla fine il risultato è stato lo stesso. No, signor Presidente. Se è vero che non è prevista una procedura aggravata in sede di Commissione, e cioè - per essere chiari - non è prevista la fase subemendativa, è altresì vero, signor Presidente, che sotto il profilo della prassi - le parlo per la 2a Commissione - ogni qual volta i relatori hanno presentato emendamenti si è sempre aperta la stagione dei subemendamenti. Quindi, se una prassi vi è stata, assolutamente consolidata, in Commissione giustizia, è stata quella di aprire la stagione dei subemendamenti ogni qual volta i relatori presentavano emendamenti. Aggiungo, signor Presidente, che, quando si è arrivati al punto della verifica del coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, e cioè quando dalla teoria - vi comunico che faremo il coordinamento - si è passati alla pratica, sia il senatore Caliendo che io abbiamo detto che non accettavamo quelle modifiche come coordinamento formale e pretendevamo che si passasse alla stagione degli emendamenti. Signor Presidente, non conosco tutti i precedenti che sono stati citati dal presidente D'Ascola. Ma, siccome uno riguarda il periodo della mia Presidenza, mi permetto di consigliarle di leggere il Resoconto di quella seduta, nell'ambito del quale lei troverà scritto "all'unanimità dei presenti". E, quindi, non vi è stato alcun contrasto in ordine al passaggio alla sede del coordinamento. Lei comprende che non è una differenza di poco conto. E ho detto detto questo per una forma di precisione in generale. Aggiungo, signor Presidente, una piccola annotazione sul coordinamento: lei ha letto l'articolo 103 giustamente ha fatto riferimento all'errore materiale, poi al coordinamento meramente formale e al contrasto con altre disposizioni. Ebbene, non è scritto da nessuna parte che una Commissione deve accedere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Una Commissione può tranquillamente venire in Aula e addirittura votare un provvedimento in contrasto con il parere della Commissione bilancio e l'organo di garanzia della correttezza del procedimento legislativo è il Presidente della Repubblica, che può rinviare il deliberato alla Camera con un suo messaggio. Dico questo perché affermare che il coordinamento è automatico sulla base delle condizioni poste dalla Commissione bilancio significa dire che la Commissione bilancio ha la capacità di modificare i testi per tutte le Commissioni di questo Senato. E ciò evidentemente, signor Presidente, non mi pare in linea con il Regolamento. Dopo di che il Presidente Zanda ha detto che è un provvedimento strategico che gli esponenti del Partito Democratico vogliano e intendano chiudere in questa legislatura. Sono d'accordo con voi.

si risolverebbe non in un provvedimento strategico, ma nell'ennesimo strategico *spot* propagandistico preelettorale.

il concorso di tante volontà e il contributo importante venuto da tante parti per la definizione del testo. Mi riferisco anche al contributo

che lo renderebbero quindi debole rispetto all'intento - che mi pare invece assolutamente condiviso - di farne uno strumento forte, che segna una svolta importante nell'ordinamento in termini non solo alle organizzazioni criminali, ma anche a fenomeni gravissimi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione e di soggezione di pezzi - speriamo il più possibilmente rari - della pubblica amministrazione al volere di interessi illeciti, talvolta organizzati anche criminalmente. Credo che questa fragilità non esista, e non soltanto per le ragioni che sono state qui dette e per il principio citato dal presidente D'Ascola, ma anche per un motivo che attiene molto più semplicemente al valore e al peso del

volevo dire, perché francamente mi dispiacerebbe e troverei ingiusto, per il lavoro fatto e per l'intenzione politica versata in questo provvedimento, che una discussione di natura procedurale possa mettere in dubbio l'intenzione, la volontà e la forza che nel disegno di legge si sono espresse da parte delle diverse forze parlamentari.

il voto sulla questione pregiudiziale è stato così evidente e le ragioni poste a sostegno della questione sospensiva sono sostanzialmente identiche

è stata rivendicata come un grande antidoto al terrorismo. La musica e le arti sono il migliore deterrente nei confronti della cultura della paura

«Progetto scuola inCanto» di Roma, ancora una volta a testimonianza di quanto questi linguaggi possano aiutare tutti. E lo diciamo da

potranno contrastare l'omologazione del *web* e rendere estetico ciò che oggi è anestetizzante.

Signora Presidente, come è noto, nella serata del 3 giugno Torino è stata colpita da un da un grave incidente legato alla finale di Champions League, che si svolgeva in Scozia. Le attività parlamentari momento e non c'è stata, quindi, occasione di fare una comunicazione al riguardo. È noto a tutti che purtroppo, nei giorni scorsi, è deceduta Erika, una delle ragazze ferite. Il mio intervento vuole sottolineare che, dopo quegli accadimenti, nella serata di ieri a Torino c'è stata purtroppo un'ulteriore coda legata agli avvenimenti di piazza San Carlo, seppur indirettamente. Dopo quegli avvenimenti il sindaco di Torino, in accordo con il prefetto e il questore, ha scelto di emanare una serie di direttive più rigide

in qualche forza politica, l'idea che la colpa di far rispettare le norme, volute peraltro dal sindaco di Torino e che noi sosteniamo fino a quando saranno in vigore - possa ricadere sulle Forze dell'ordine e non sul teppismo politico del centro sociale. Credo sia utile che questa comunicazione venga trasmessa anche al Ministro dell'interno e doveroso portare la solidarietà alle Forze dell'ordine. Rivolgo poi un invito all'amministrazione di Torino a proseguire sulla strada della legalità, così come è stata intrapresa.